dopo un lungo periodo di gestazione, durato tanti mesi, questo provvedimento arriva oggi in Aula, e mi auguro possa essere anche licenziato.

Credo che tutto questo sia stato fatto, per quanto possibile. Mi auguro quindi che oggi, anche di fronte all'accoglimento di molti emendamenti, e anche di fronte ad altri emendamenti che ho presentato,

un provvedimento cardine per noi italiani all'estero. L'Atto Senato n. 1460 alla vostra attenzione, infatti, incide profondamente su ben due delle tre rappresentanze elettive della cosiddetta altra Italia, all'interno delle istituzioni della Repubblica italiana: i COMITES (Comitati degli italiani all'estero) ed il CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero). Quando si dice altra Italia, mi si permetta di ricordare, ci si riferisce ad un popolo di quasi 4,5 milioni di cittadini ufficialmente registrati nell'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, una popolazione in continua crescita con una maggioranza di persone la cui età è inferiore ai quarant'anni ma che, di fatto, sono una piccola frazione delle decine di milioni di italiani e discendenti di italiani che effettivamente risiedono all'estero. Per inciso, mi si permetta con l'occasione di segnalare a chi di dovere che proprio in conseguenza di ciò il totale della popolazione dei cittadini italiani non è di oltre 60 milioni, come viene universalmente indicato, specie sulla stampa, ma di circa 65 milioni. Si tratta dunque di un momento parlamentare molto importante per noi e molto sentito dalle nostre comunità all'estero. In occasione del precedente approdo in Assemblea, avevamo già ricordato brevemente la *ratio* storica sottostante a queste specifiche disposizioni legislative. Il nostro Paese è stato protagonista nella sua storia contemporanea di un fenomeno migratorio senza eguali al mondo sia per quantità, che per durata

e andando in ogni parte del mondo. Nessun altro Paese al mondo ha vissuto un simile fenomeno. Comune denominatore di tante diverse esperienze migratorie sono stati due fattori: primo, il bisogno di partire; secondo, la pressoché totale mancanza di considerazione da parte dello Stato. A porre fine a questo secondo aspetto, indegno della storia e della cultura dell'Italia, sono finalmente intervenute le disposizioni legislative che hanno riconosciuto ed istituzionalizzato la presenza degli italiani all'estero: la legge n. 205 del 1985, istitutiva dei COMITES (e successive modificazioni); la legge n. 386 del 1989 (e successive modificazioni), istitutiva del CGIE; le leggi costituzionali n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001 sulla circoscrizione Estero e la legge n. 459 del 2001, la cosiddetta legge Tremaglia, sulla disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Principio cardine di tutti questi provvedimenti legislativi è il riconoscimento della consequenzialità dei diritti politici e di elettorato attivo e passivo al possesso della cittadinanza italiana. Non si consegue il diritto-dovere in ragione del censo o di quante tasse si pagano; non sulla base della conoscenza della società o della politica italiana (chi potrebbe decidere non sulla base del sesso, della religione o della residenza. All'estero, come in Italia, è solo l'essere cittadini italiani che dà diritto all'elettorato attivo e passivo. Si badi - per inciso - che per molti italiani emigrati all'estero non è stato facile conservare la cittadinanza e, quindi, se lo hanno fatto (in un certo senso) hanno meritato ancora di più di poter dire la loro sull'organizzazione ed il progetto politico della madrepatria, a prescindere da dove risiedono. per quanto riguarda le rappresentanze cosiddette di base degli italiani all'estero (ovvero i COMITES), grazie alla meritoria opera di raccordo del relatore collega senatore Tofani (che noi italiani all'estero non possiamo che ringraziare, sentitamente, per aver posto la sua pazienza, capacità ed autorevolezza al servizio della nostra causa), vengono introdotti nell'ordinamento italiano alcuni opportuni aggiornamenti che razionalizzano il settore e mettono le migliori premesse

appare opportuno mettere in evidenza che: si riduce di un terzo (da 90 a 60) il numero dei COMITES sul territorio della circoscrizione Estero; si assicura un premio di maggioranza alla lista vincitrice del COMITES; si aboliscono gli oltre 30 rappresentanti non elettivi del CGIE; si introduce un Consiglio generale degli italiani nel mondo, nel quale sono presenti, come doverosamente richiesto da noi diverse volte, i rappresentanti delle Regioni. A tale riguardo, appare a noi particolarmente benemerito il fatto di aver posto come discrimine generale della nuova normativa il criterio della selezione democratica. Il carattere elettivo delle rappresentanze degli italiani all'estero riguarda infatti sia i livelli di base che quelli massimi. infatti, data la stessa origine elettorale e la stessa tecnica di selezione, sono solo i *quorum* di successo elettorale a distinguere i consiglieri COMITES dai parlamentari eletti *ex lege* n. 459 del 2001. non riguardava invece *in toto* il livello intermedio del CGIE, nella cui composizione attuale oltre un terzo dei componenti non sono eletti (bensì nominati), ma l'Atto Senato n. 1460, attualmente all'esame, limita i nominati ai soli rappresentanti di Regioni e Province autonome ed ai presidenti di ANCI e UPI (Associazione nazionale dei Comuni italiani e Unione delle Province italiane) e dunque rispristina il principio elettivo tanto democraticamente caro a noi italiani all'estero anche nel CGIE. Non è cosa da poco. La natura democratico-elettiva di questi enti, regolati da leggi dello Stato italiano ed in tutto titolati a fregiarsi del rango di istituzioni della Repubblica è, infatti, talmente forte da legittimarli anche al di fuori dei confini sovrani dello Stato e della legislazione italiana. Al riguardo, è bene che non sfugga a nessuno - e per questo ritengo sia importante ribadirlo qui, nella Camera alta che, a differenza delle rappresentanze diplomatico-consolari che costituiscono propaggini statuali all'estero tradizionalmente riconosciute dal diritto internazionale, le rappresentanze COMITES sono in realtà accettate all'interno di sistemi sovrani terzi rispetto al nostro, solo in quanto ritenute degne e compatibili con i locali criteri giuridici di rappresentanza democratica di interessi collettivi e legittimi. Vorrei tornare su un punto, cosciente di trovarmi di fronte ad una posizione personale non ancora suffragata dalla dottrina o dalla giurisprudenza, ma intento a fare la mia parte *de iure condendo*. La proiezione del vigore legislativo italiano in ambiti giuridico-territoriali esclusi dalla nostra sovranità (cioè tutti quelli della cosiddetta circoscrizione Estero) non sarebbe possibile se ivi non si riconoscesse - più o meno esplicitamente - la coerenza di tali dispositivi con i locali principi di gestione democratica della *res publica.* I COMITES, illustri colleghi, non sono e non saranno mai un mero consesso consultivo del Ministero degli affari esteri. Non lo sono per la legge italiana e non lo sono per le autorità dei luoghi nei quali esplicano la loro meritoria attività. Sono molto più importanti, per fortuna! Ho citato, al riguardo già in passato, alcuni esempi tratti dalla recente attività politica sul territorio della circoscrizione Estero. Diversi Diversi *Laender* tedeschi - oltre a consentire l'esistenza dei COMITES italiani sul loro territorio - considerano i vertici da loro selezionati democraticamente (i cosiddetti Inter comites) come i legittimi interlocutori istituzionali con le comunità italiane ivi residenti. Ai fini della gestione della locale *res publica* sono loro - e non l'ambasciatore rappresentante del Governo italiano a Berlino - a rappresentare gli italiani ivi residenti, perché anche secondo la legge tedesca quelle rappresentanze locali sarebbero selezionate con quelle stesse procedure democratiche. In Svizzera, di recente, in seguito all'attività di *lobbying* politica esercitata dai COMITES locali, il cantone di San Gallo è tornato indietro sulla decisione di tagliare i fondi per i corsi di lingua italiana, riconoscendo (per gli stessi motivi sopra detti) a quegli interlocutori istituiti con legge italiana la dignità di rappresentanza di interessi locali svizzeri. Ecco dunque perché il criterio di elezione democratica è talmente è talmente importante. Ecco perché noi italiani all'estero siamo fieri che esso informi di sé ogni nostra istituzione. Ed ecco perché il sistema istituito dal legislatore italiano può trovare piena applicazione anche all'estero. Sulla base di queste considerazioni,

Noi invece parliamo di una legge che dovrà trovare applicazione in tutto il mondo e che dovrebbe rispondere alle esigenze delle nostre comunità che vivono in tutti i Paesi del mondo. Questi Comitati, e il Consiglio generale degli italiani all'estero, hanno svolto un ruolo estremamente importante in questi vent'anni di storia, però, oggi dobbiamo prendere atto della profonda trasformazione degli italiani all'estero e della composizione della nostra comunità.

Questi organismi, eletti a suffragio universale, devono essere i veri interlocutori dei parlamentari, strumenti indispensabili se vogliamo compiere il nostro lavoro di rappresentanza di collegi cui apparteniamo io ed il collega Fantetti conta oltre 60 Nazioni, ed è impensabile che un senatore possa conoscere tutte queste realtà e possa avere la capacità di fare sintesi dei bisogni di una Nazione. Questi organismi hanno un vantaggio nei confronti di tutte le altre associazioni o organizzazioni di partito: sono il risultato di un'elezione democratica e, dunque, chiamati a fare sintesi. Questo è estremamente importante per il nostro lavoro, come lo è il Consiglio generale, un luogo indispensabile per fare sintesi della politica generale che bisogna sviluppare per gli italiani all'estero.

enti, istituzioni e associazioni storiche, che sono state importantissime per la storia degli italiani all'estero poiché hanno costruito la storia dell'integrazione degli italiani nel mondo.

consiglieri del Consiglio generale degli italiani all'estero che verranno a Roma per svolgere il loro lavoro siederanno a un tavolo alla presenza dei vari rappresentanti dei Ministeri di competenza, quindi con lo Stato centrale, e allo stesso livello degli assessori regionali.

il Governo e il relatore possano accogliere gran parte degli emendamenti da noi presentati, che vanno in direzione di rafforzare il ruolo politico e istituzionale della rappresentanza degli italiani all'estero, perché credo che sia

che nell'interesse degli italiani all'estero. Mi auguro anche che questo dibattito serva a far capire ai partiti che è importante

impegnare in questo collegio come farebbero per qualsiasi altra Regione, e non vederlo con gli occhi della nostalgia. La nostalgia non fa più parte dei dei sentimenti degli italiani all'estero: i nostri figli nati all'estero hanno un legame profondo con l'Italia, un legame culturale, di valore, non nostalgico, e desiderano dare un contributo all'Italia. Questo si tenta di fare con la presente riforma, e mi auguro pertanto che vengano accolti gli emendamenti migliorativi.

in materia di riforma dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero, elaborato dalla Commissione affari esteri trasmesso all'Assemblea e, successivamente, rinviato per un ulteriore approfondimento alla Commissione, che ha dato un nuovo mandato a riferire in Aula, è sicuramente un compromesso possibile tra le forze politiche di fronte a un problema diffuso in tutto il mondo che presenta problemi difficilmente risolvibili. La proposta normativa fatta propria dalla maggioranza ridisegna l'articolazione territoriale dei COMITES, ridefinendone i compiti e la composizione. riguarda il Consiglio generale degli italiani all'estero, si prevede l'appartenenza di diritto dei presidenti degli Intercomites, superando un'inopportuna incompatibilità nella duplice appartenenza ai suddetti organismi di rappresentanza delle comunità italiane nel mondo. Viene invece eliminata la componente di nomina governativa, la cui soppressione ha suscitato forti dissensi nell'articolato mondo dell'associazionismo. Credo però che la presenza degli assessori regionali all'emigrazione sia un fatto certamente positivo, perché consente una partecipazione diretta delle Regioni che finanziano a vario titolo tante manifestazioni culturali che vengono organizzate durante l'anno. Di conseguenza, è giusto che ci sia questa integrazione e che si risponda direttamente alle iniziative che vengono proposte, anche se, a mio avviso,

verso l'estero, ma chi è lontano dalla madrepatria si sente un italiano integrato al cento e non riesce a vedere le divisioni che ci possono essere nell'ambito della nostra organizzazione nazionale. Un'ulteriore e fondamentale novità è quella dell'inclusione delle rappresentanze delle autonomie locali e regionali. Questi sono i tratti salienti della riforma, rispetto alla quale sono presentatore di talune proposte di modifica, che mi sembra non siano state accettate. Alcuni dei miei emendamenti al testo unificato propongono il superamento del sistema del voto per corrispondenza e l'istituzione del voto nei seggi elettorali anche al di fuori dei confini nazionali. Ma chi può essere soddisfatto di come sono andate le cose per il voto degli italiani all'estero? Tutta la stampa ha parlato di *vulnus* che ci sono stati nel sistema di voto degli equivoci che si sono posti all'attenzione di coloro i quali hanno partecipato al voto. Mi rendo tuttavia conto che è difficile organizzare un voto nelle cabine elettorali,

il dibattito svolto in Commissione non ha trovato una soluzione adeguata di cui purtroppo ci sarebbe molto bisogno. la reintroduzione di una limitata rappresentanza di consiglieri del CGIE di nomina governativa, venendo incontro alle istanze del mondo delle associazioni e dei patronati, la presenza nel CGIE della rappresentanza delle Camere di commercio italiane nel mondo, per il significato e il ruolo assunto nel corso degli anni.

con tantissimi connazionali che hanno fatto cose importantissime, ponendosi all'attenzione degli Stati in cui essi vivono, ma anche al di fuori dei confini di quegli stessi Stati.

la ridefinizione del sistema di partecipazione degli enti locali e regionali. Le Regioni, in particolare, alla stessa stregua degli enti locali, devono assicurare nel CGIE la loro rappresentanza, attraverso la Conferenza delle Regioni, finalizzata a garantire nei confronti dei nostri connazionali all'estero una tempestiva sintesi politico-amministrativa necessaria ad indirizzi legislativi armonici tra loro. La realtà però

Penso che la concezione in qualche modo sia rimasta lontana dal cambiamento che c'è stato nel corso degli anni. In qualità di Presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, mi sono disposto in più occasioni

vada dunque approvato nel più breve tempo possibile, per dare quelle risposte che gran parte degli italiani all'estero aspettano da noi.

come sempre, caratterizzano l'approccio di questa maggioranza in ogni occasione, oggi in particolare relativamente ad una materia importante come quella della rappresentanza degli italiani all'estero. Qualcuno potrà ironizzare

rappresentando la cultura, la lingua e quanto di meglio dovrebbe uscire da questi comitati.

vanno ai COMITES o al CGIE, che servono per rappresentare una cultura. Ecco allora perché dobbiamo riflettere su come andare avanti con questa legge,

buona, una legge di rappresentanza vera, con la R maiuscola.

non voglio neppure essere ripetitivo, in quanto la relazione del senatore Tofani è stata precisa, puntuale e dettagliata. Evidentemente il testo oggi regolamenta i COMITES e il

di fare i complimenti non solo ai colleghi parlamentari, ma anche agli uffici che hanno sostenuto questo impegno. La disciplina attualmente in vigore necessita di una riforma e di un riassetto, soprattutto alla luce della rilevante novità costituita dall'introduzione, come si è più volte ribadito, del diritto di voto per i nostri cittadini residenti all'estero e la previsione di parlamentari eletti nella circoscrizione

È necessario procedere a questa riforma allo scopo di consentire il rinnovo degli organismi prima citati secondo le nuove e più idonee modalità. Nel Testo unico vengono modificate le soglie minime di consistenza delle collettività italiane nel mondo necessarie per procedere alla formazione di detti organismi. Comitato è chiamato a redigere una relazione annuale per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Viene, inoltre, stabilito che deve essere istituito un Comitato dei presidenti, detto Intercomites, quando in un Paese viene formato più di un Comitato.

secondo il testo proposto, andrebbe modificata la sua denominazione in Consiglio degli italiani all'estero, e avrebbe 82 membri; ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites, o gli assessori con delega all'immigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani e dell'Unione delle Province d'Italia.

nel processo di sviluppo della partecipazione attiva nella vita politica da parte delle collettività italiane nel mondo e allo stesso tempo costituiscono l'organismo essenziale per il collegamento permanente con il nostro Paese e le sue istituzioni. Sebbene siano di basilare importanza, è d'obbligo ricordare che le attuali strutture andrebbero rinnovate, come appunto ricordavo all'inizio, in quanto potrebbero essere causa di duplicazione anche delle proprie funzioni. Ciò comporterebbe evidentemente inefficienza a livello burocratico e conseguentemente spese esose e anche inutili.

nel corso dell'esame degli emendamenti tutte le proposte e i contributi della Lega Nord siano accettati, anche attraverso eventuali riformulazioni, purché la sostanza resti la stessa.

all'esame dell'Aula era atteso dai cittadini italiani nel mondo (circa 4 milioni di elettori), anche perché la scadenza naturale per il rinnovo dei rappresentanti di questi organismi era prevista nel 2009.

Il COMITES (organismo istituito in base alla legge 8 maggio 1985, n. 205) è concepito come punto di riferimento diretto della comunità italiana residente nella circoscrizione consolare. Con l'avvento dell'elezione dei 18 parlamentari eletti all'estero, molte cose sono cambiate nel mondo dell'emigrazione italiana, anche se si tende a trascurare l'importanza dei rappresentanti all'estero e del conseguente impatto sull'intero sistema delle rappresentanze delle nostre comunità, così come risulta dalla vigente normativa in tema di COMITES e di CGIE. Bisogna prendere atto di questa nuova realtà: è anche, e soprattutto, per questi motivi, che una riforma dei due organismi era diventata necessaria. Credo che il COMITES, come riformato oggi con questo provvedimento, abbia un ruolo ancora maggiore nelle relazioni delle nostre comunità all'estero, soprattutto se riuscirà a dare spazio ai giovani e a quanti desiderano impegnarsi nel mondo dell'emigrazione per avvicinare sempre più i nostri concittadini all'estero alla madrepatria, al nostro bel Paese. Il CGIE, l'organismo fondato il 6 novembre 1989 con il ruolo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso il Governo e le autorità politiche, è anche punto di raccordo tra COMITES e parlamentari della circoscrizione Estero. Ora, dopo l'elezione dei 18 parlamentari all'estero, avvenuta per la prima volta nell'aprile del 2006, la funzione del CGIE di fatto è in parte cambiata. Quindi, oggi il ruolo del CGIE non è più quello originario, che risale alla sua fondazione, perché molte incombenze e funzioni sono automaticamente passate di fatto ai parlamentari della circoscrizione Estero. Oggi non si può perpetuare il carattere inutilmente assembleare di tale organismo, che comporta un dispendio di tempo impiegato in dibattiti spesso sterili anche perché viziati da visioni eccessivamente di parte; vengono invece, del tutto trascurati gli aspetti operativi della sua attività, quali iniziative concrete a favore di gruppi delle nostre collettività, borse di studio, scambi e contatti con gruppi in Italia, formazione professionale. In tal modo tutte le risorse disponibili risultano impiegate solo per le spese di gestione - ed il caso del CGIE è evidente - con la pletora di riunioni, delibere, atti di indirizzo, assunzione di esperti, indagini conoscitive, come se i membri non venissero già dall'estero. Ed è questo un sintomo eloquente della concezione "grandiosa" che si ha del CGIE, nato del resto sul modello francese. Ad esempio, la proposta di Presidenza, l'invio di documenti vari, relazioni, programmi, pareri, che la proposta stessa prevede numerosi, mentre mancano da questo quadro iniziative concrete che vadano a beneficio delle nostre comunità, del loro sviluppo reale, soprattutto dei loro legami con l'Italia e dei rapporti, anche economici, con le sue numerose e varie espressioni produttive ed imprenditoriali. In conclusione, signor Presidente, mentre ritengo che il COMITES sia un organismo necessario per le comunità italiane nel mondo perché più vicino al cittadino e alle sue problematiche ed aspirazioni penso che, il CGIE, secondo ciò che abbiamo visto negli ultimi anni, e soprattutto ultimamente in vari convegni (da ultimo a Torino), vada rivisto e riformato profondamente. Mi auguro, quindi, che questo disegno di legge venga approvato ed in seconda lettura alla Camera si possa trovare un consenso *bipartisan* ancor più vasto per poter dare al CGIE un ruolo più consono alla luce delle esperienze del passato e soprattutto della nuova realtà odierna. Mi dispiacerebbe se si dovesse arrivare un giorno a dar ragione a quanti pensano e suggeriscono, non ultimo l'*ex* Ministro degli affari

Fermi restando gli argomenti già previsti per questa settimana, la seduta di sindacato ispettivo, già prevista per le ore 9,30 di giovedì, è posticipata alle ore 15. La prossima settimana, in vista delle manifestazioni programmate per la festa della Repubblica, 1'Assemblea terrà seduta nella giornata di mercoledì 1° giugno, con all'ordine del giorno i disegni di legge recanti rispettivamente proroga termini in materia di federalismo fiscale e giornata della memoria per le vittime dei disastri ambientali e industriali, nonché le mozioni Ramponi sulla sicurezza da minaccia cibernetica e Biondelli sul problema dell'autismo. È stato infine stabilito che nella seduta del 7 giugno prossimo il Senato commemorerà la figura di Cavour, in occasione del 150° anniversario

*relatore*. Signor Presidente, la mia sarà una replica molto breve, anche perché abbiamo avuto già modo di intervenire su questo tema

in questa fattispecie sono quantomeno ingenerose o frutto della non conoscenza del testo, perché non abbiamo fatto né un copia e incolla, né le altre cose che lei, senatore Pedica, ha detto. Posso capire che si dissenta, perché

da me interpretato probabilmente in modo non adeguato o addirittura erroneo, comunque mi ha portato a pensare che verosimilmente lei condividesse quelle cose.

voglio solo dire con grande rispetto che questo è un lavoro nato in Parlamento e voluto dai parlamentari. Il Governo non ha presentato, volutamente, alcuna proposta di riforma e ha solo accompagnato il dibattito, certamente intenso, che si è svolto prima nel Comitato ristretto e poi in Commissione. Il ringraziamento va quindi al presidente Dini e a tutti i membri della Commissione, oltre ovviamente a chi è stato protagonista di questa vicenda. Vorrei aggiungere una questione quasi personale, perché non è facile per uno come me, che ha vissuto una vita politica insieme all'onorevole Tremaglia, trovarsi oggi ad affrontare un tema che sembra, da un certo punto di vista, contrastare con l'architettura di quello che è stato per me anche un maestro. Credo invece che, che, proprio nel rispetto di quella continuità di pensiero, oggi stiamo procedendo ad un momento di grande rilevanza, che si allinea con quelli che sono stati il pensiero e l'azione dell'onorevole Tremaglia. Quando sono stati creati, con una riforma costituzionale, i parlamentari italiani eletti all'estero, si è ottenuto un risultato credo storico all'interno di questo Parlamento, ma nello stesso momento era evidente che una struttura come quella del CGIE, che per anni aveva svolto un compito fondamentale, assimilabile a quello di un piccolo Parlamento a lato del Parlamento vero, perché lì non c'erano i rappresentanti degli italiani nel mondo, andava in qualche modo ricollegata

nel senso che quella cultura, che portò il CGIE ad essere rappresentanza degli italiani nel mondo ed interlocutore del Governo, non c'è più. Vogliamo cambiargli il nome per non creare problemi? Non ho francamente, su queste cose, nessuna crociata da fare. invece creato un elemento che oggi è importante, anche con la riforma del Titolo V. Oggi le Regioni, anche nel rapporto con le proprie comunità all'estero,

discutono delle politiche regionali, che riguardano anche fondi e politiche di assistenza sociale e sanitaria, e insieme elaborano una politica per gli italiani all'estero

che questa posizione feroce di opposizione sia legata al fatto più evidente che non ci sono più membri del CGIE eletti dai partiti. Credo sia un grande risultato, e penso che il CGIE debba essere formato dagli italiani e dalle Regioni, perché questo è il loro interesse, e che i funzionari degli italiani eletti all'estero oggi non abbiano più ragione di essere di diritto rappresentati. Siccome sono aperti i COMITES (li abbiamo anche allargati), credo che dalla base possano benissimo presentarsi tutti,

parere non ostativo, con l'occasione segnalando, quanto all'emendamento 7.206, che la disposizione, agendo sui mandati elettorali in corso, potrebbe comportare un'irragionevole disparità di trattamento».

Esprime inoltre parere non ostativo sulle proposte parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.1 (testo 2), 1.7, 1.206,

1.218, 1.5, 1.219, 2.201, 2.202, 2.3, 2.1 (testo 2), 2.2, 2.5, 3.201, 3.202, 3.203, 4.201, 4.202, 5.202, 5.203, 6.200, 6.201, 6.203, 7.201, 7.202, 7.203, 7.204, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.205, 10.201, 10.1, 10.202,

16.201, 16.203, 16.204, 11.202, 14.203, 16.202, 22.2, 22.0.1, 24.100, 24.7,

Esprime inoltre parere non ostativo sulle proposte 12.6 e 12.205 osservando che sono suscettibili di determinare risparmi rispetto al testo in esame. Pertanto la Commissione segnala che, in caso di loro approvazione, andrebbe rideterminato, sulla base di una quantificazione da acquisire dal Governo, l'ammontare degli oneri indicati nell'articolo 23, comma 2. Esprime, altresì, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

riferimento a tutto il mondo, ma il mondo è una realtà complicata, grande e difficile. Si tratta solo di dare una possibilità in più a chi ha la responsabilità, nel caso particolare il Ministro degli affari esteri, di potere insediare in casi particolari, dove vi sono grandi comunità, più comunità, più di un Comitato. Oggi è già così, ed è già possibile avere più di un Comitato che dipenda da uno stesso ufficio consolare.

lavoratori che tornano tutte le sere in Italia.

tale. L'emendamento 2.3 vuole esplicitare la situazione che il testo approvato dalla Commissione riassume sotto la dicitura, forse troppo generica, «non è possibile procedere all'elezione dei Comitati». Noi proponiamo di individuare le cause di questa impossibilità ad indire le elezioni nella mancanza del numero minimo sufficiente di cittadini italiani e dell'impossibilità a svolgere concretamente le stesse elezioni nella distribuzione troppo ampia dei cittadini su più aree consolari.

Passiamo alla votazione

che questi Comitati abbiano la certezza di ottenere risposte da parte dell'Amministrazione.

al lavoro che compie il COMITES, soprattutto quando chiediamo a questi Comitati di valutare la qualità dei servizi che la rete consolare e i consolati danno ai nostri concittadini. Ho sentito il ministro Brunetta affermare in tutti i programmi televisivi e in tutti i giornali che i cittadini italiani devono valutare e giudicare il lavoro della propria Amministrazione. Mi sono riempito la testa di queste dichiarazioni. si chiede semplicemente che il rapporto che redige un COMITES sulla qualità dei servizi di un consolato su un territorio

Credo sia nella logica più elementare del discorso del ministro Brunetta. In detto caso si chiede di dare questo diritto non a qualsiasi cittadino, ma ad un Comitato eletto a rappresentarlo.

Perché insisto sul termine di risposta, Presidente? So che su questo abbiamo dibattuto in Comitato ristretto. Mi si dice che anche in Italia le istituzioni non hanno una garanzia di un termine di risposta.

non gestiscono infatti risorse economiche, non danno risorse economiche, ma esprimono i bisogni e le potenzialità della nostra collettività. È bene che questi Comitati abbiano la certezza di avere una risposta, perché oggi sappiamo che non

l'emendamento 4.250 arricchisce il testo uscito dalla Commissione definendo maggiormente le funzioni dei Comitati, dando loro nuove competenze, chiarendo il rapporto con le altre autorità che curano gli interessi degli italiani all'estero e stabiliscono norme di trasparenza e tracciabilità In particolare, i Comitati, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il rapporto con le autorità consolari viene rafforzato, poiché, da una parte, è compito del consolato informare le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta, nonché di rendere partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata; dall'altra parte, il Comitato può rappresentare le istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali. È da rilevare, inoltre, il fatto che, con il presente emendamento, si dà ai Comitati una funzione di consulenza normativa, ossia la possibilità di formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, nonché accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero. per quello che riguarda l'Italia dei Valori, si valorizza la competenza degli stessi maturata sul campo nel processo normativo. In sostanza, si trasferiscono ai Comitati le poche residue competenze che adesso esercita in esclusiva il CGIE per farne ancora di più il perno gravitazionale a livello locale delle multiple istanze provenienti dalle comunità degli italiani. dell'articolo 4, che si propone di emendare, che tuttavia vengono proposte le novità più rilevanti, in quanto vengono individuati meccanismi per aumentare la trasparenza e la responsabilità dei Comitati nei confronti degli elettori. Ciò si ha ponendo l'obbligo in capo all'organismo di redigere ed elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare e un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Per rendere maggiormente tracciabile l'utilizzo delle risorse affidate ai Comitati, nell'emendamento si prevede che alla relazione siano allegati il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo di cui all'articolo 6 del testo della Commissione. Quindi, il Ministro degli affari esteri invia il documento unico, acquisendone i relativi pareri, ai seguenti destinatari:

sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Infine, il documento unico viene presentato dal Ministro al Parlamento aprendo un dibattito pubblico per valutare gli eventi dell'anno precedente e tracciare prospettive e indirizzi per il triennio successivo. In definitiva, l'emendamento in questione, trasferendo le competenze esercitate dal CGIE ai Comitati, consegue l'obiettivo di semplificare e rendere efficiente il panorama generale delle forme e degli istituti di rappresentanza degli italiani all'estero, promuovendo così una più efficace tutela dei loro interessi e dei loro diritti.

In fine al comma 8 si aggiungerebbe il seguente periodo: «Un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente». Al comma 9 la parola «e» sarebbe sostituita dalle parole: «al Presidente dell'Intercomites del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero dello stesso Paese,». Infine, al comma 11 sono inserite le parole: «cui la stessa darà riscontro», ma senza specificare i tempi. i vari emendamenti che su questo tema sono stati presentati dal senatore Micheloni. L'unico punto che non posso accettare è quello dei tempi, anche perché credo che qualora non vi fossero dei tempi adeguati, anche grazie alla presenza dei parlamentari eletti nelle circoscrizioni Estero ci sarebbero tutti gli strumenti per poter fare in modo che vanga effettivamente

l'emendamento 5.200 sopprime l'istituto degli Intercomites, poiché, come si evince dal disegno di legge a mia firma e dagli emendamenti sinora illustrati, la *ratio* della proposta di riforma dell'Italia dei Valori è quella di stabilire un dialogo diretto tra le comunità italiane all'estero e i rappresentanti centrali, tramite l'unica intermediazione esercitata dai Comitati. Sono questi, infatti, e non forme ulteriori di aggregazione, come gli Intercomites e il CGIE, che si relazionano ai consolati, ai parlamentari eletti all'estero, al Ministero degli affari esteri e al Parlamento nel complesso. La ragione di creare tale filo diretto risiede sia nella volontà di risparmiare risorse tagliando istituiti ormai pleonastici, sia in quella di veicolare meglio le istanze di cittadini italiani all'estero, senza che interessi mediati e forme di potere acquisite, come si generano spesso anche nel CGIE, possano influenzarle. I COMITES, infatti, sono più vicini alla popolazione, poiché composti da membri eletti direttamente dagli italiani all'estero in ciascuna circoscrizione consolare e, quindi, risultano più titolati ad esprimere genuinamente problemi e proposte dei nostri connazionali espatriati.

tende ad evitare che si concentrino troppe funzioni su una sola persona. Non dimentichiamo mai che queste istituzioni istituzioni che stiamo rinnovando, che siano COMITES o CGIE, sono composte da persone elette a cariche importanti per la comunità, ma a titolo assolutamente gratuito: fanno del volontariato. Qui non stiamo mettendo in piedi delle strutture

appare necessario evitare di concentrare troppe funzioni sulle stesse persone. Questo è l'obiettivo dell'emendamento 5.7.

è d'accordo sulla riformulazione che ho letto, ovviamente aggiungendo il termine temporale di 180 giorni.

ovviamente prendo atto di quanto lei ha dichiarato, anche se i contenuti della riformulazione non evocano assolutamente necessità di coperture;

4.206 non sembrano assolutamente comportare oneri, per cui è possibile dare subito un parere di nulla osta.

sulla base dell'esperienza vissuta anche in questa legislatura, va a porre rimedio ad eventuali forzature. Pertanto, è particolarmente raccomandabile.

che chiarisce il rapporto tra le autorità consolari e i COMITES, giacché non tutte le funzioni possono essere concentrate sulle autorità consolari. Occorre sentire i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero del Paese di competenza.

parere è conforme a quello del relatore.

So bene che ogni volta che parliamo di voto per corrispondenza nel Parlamento italiano si parte dal presupposto che non è un sistema sicuro, ma altri Paesi europei il voto per corrispondenza è una realtà.

senatore Firrarello.

che sostituire il voto per corrispondenza, come previsto nell'emendamento 12.205 - so che l'articolo 12 è stato accantonato, ma anticipo la questione, che potrei risolvere ritirando l'emendamento

individuare una soluzione, che è già inserita negli emendamenti 14.2 e 14.3, magari attraverso una

*«*Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, devono essere verificate la corrispondenza del documento d'identità, inserito dall'elettore nella busta contenente il tagliando, con il nominativo risultante dagli elenchi consolari,

Sono d'accordo con il relatore e apprezzo anche che abbia seguito il modello spagnolo e non quello svizzero, che in Italia è difficilmente applicabile.

senatore Firrarello a ritirare

All'articolo 16, il comma 4 e riformulato come segue: «Se uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente nomina scrutatore uno degli elettori. Se il Presidente è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina del sostituto».

18.204 è estremamente importante perché con l'articolo 18 si modifica il sistema di voto, che attualmente è proporzionale puro.

L'ho detto all'inizio: questa legge riforma qualcosa di esistente all'interno di due voci di spesa del Ministero degli affari esteri che hanno subito tutti i tagli come tutti gli altri capitoli, e non si creano spese si deve fare con quello che c'è. Ricordo che stiamo parlando di organismi di volontariato.

appare, ad avviso dell'Italia dei Valori, come un ente pleonastico, stante le recenti modifiche istituzionali apportate alle forme di rappresentanza e considerate le mutazioni occorse al fenomeno dell'emigrazione. Le principali ragioni che ci inducono a sostenere che, per molti aspetti, le funzioni assegnate al CGIE nel 1989 sono ormai state assunte da altri organismi di rappresentanza sono l'istituzione della circoscrizione Estero e l'elezione dei rappresentanti parlamentari dei cittadini italiani residenti all'estero, disciplinata dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459. attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero è la manifestazione del principio costituzionale espresso dall'articolo 67 della nostra Costituzione (che recita: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»), in quanto individua nel parlamentare in genere - ed in quello eletto nella circoscrizione Estero in specie il «rappresentante *erga omnes*» delle comunità italiane radicate fuori dai nostri confini. In particolare, con la creazione della circoscrizione Estero, vengono ad essere assorbite tutte quelle funzioni di "consulenza" del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero, le quali, a seguito della riforma elettorale, appaiono realizzate dalla figura del parlamentare. Per ciò che concerne invece le altre funzioni che la legge 6 novembre 1989, n. 368 affida al CGIE, ossia le competenze maggiormente finalizzate allo sviluppo delle potenzialità a livello locale delle comunità italiane nel mondo e delle loro risorse economiche, culturali e sociali, osservo che le stesse esigenze locali possono essere portate avanti con maggiore incisività ed efficienza dall'altro organo rappresentativo presente, ossia i Comitati degli italiani all'estero, Pertanto, con la soppressione del CGIE ed il precedente trasferimento delle competenze esercitate in esclusiva ai Comitati, quel che si vuole creare - vogliamo spiegare ai colleghi - è una rappresentanza imperniata a livello locale sui Comitati e sui consolati, con un forte dialogo programmatico fra loro, e a livello centrale sul Ministero degli affari esteri e sui parlamentari eletti all'estero. Ecco cosa vogliamo intendere con questo emendamento. In tale quadro, le riunioni generali del CGIE, di carattere meramente discorsivo e poco sostanziale, in quanto organismo composto da ben 82 membri, con cadenza pari a solo due riunioni l'anno e senza poteri vincolanti, perdono significato e senso, e l'abolizione delle stesse, non togliendo niente alla rappresentanza, reca invece un sensibile risparmio economico, che il Ministero può utilizzare per iniziative concrete in favore degli italiani all'estero. Il presente emendamento, dunque, non deve essere letto come isolato, ma in combinato con i precedenti. Pertanto, voglio precisare, che non è «una semplice cancellazione» quella che si propone, ma è una riforma complessiva dì tutto il panorama della rappresentanza degli italiani all'estero. Questo sforzo riformatore mi sembra doveroso, sia nei confronti dei cittadini all'estero, sia per ciò che attiene l'uso delle risorse pubbliche, le quali, in tempo di crisi, devono essere impiegate là dove possono effettivamente perseguire il bene pubblico con i maggiori risultati. Noi dell'Italia dei Valori vogliamo che chi guarda da lontano all'Italia sia orgoglioso di esserne cittadino, e si senta, anche all'estero, comunque partecipe di una Nazione che sa perseguire il bene non solo di chi risiede sul suo territorio ma anche di chi ne fa parte per diritto. E - concludo, signora Presidente - tutto ciò lo si ottiene soltanto disegnando un quadro efficiente, volto al risparmio, agevole e capace di stabilire un dialogo permanente fra comitati di base, consolati, parlamentari e Ministro degli affari esteri, così come proposto prima con il mio disegno di legge e ora con gli emendamenti in questione.

mi accorgo con notevole fatica, di mettere in piedi, ha poco a che vedere con l'organismo che siamo abituati ad avere oggi, ed è uno strumento che non è in contraddizione con la presenza dei parlamentari italiani del collegio Estero, uno strumento indispensabile, se vogliamo che questi parlamentari rappresentino veramente le nostre comunità che stanno all'estero e non rappresentino altri interessi di enti o strutture italiane. Questo è il fondo del problema. I parlamentari della circoscrizione Estero non sono dei tuttologi: come potete come potete immaginare che un solo parlamentare sia in grado di fare sintesi delle realtà di 60 Nazioni? Facciamo un discorso di buon senso: non è immaginabile poter

Comitato ristretto) è che diventano interlocutori non di parte dei parlamentari, ma diventano interlocutori eletti dai cittadini italiani e dunque si confrontano con i parlamentari e danno l'indirizzo alle politiche necessarie.

che il Parlamento esamini la relazione annuale del Consiglio generale degli italiani all'estero. Può sembrare che si voglia dare un ordine al Parlamento o chissà cosa; non è così. Oramai sono cinque anni che sono in quest'Aula

e potrebbe anche essere interessante un discorso del genere se non avessimo 18 parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, che in effetti hanno questo ruolo e quindi, possono svolgere ogni azione, tant'è vero che anche qui

Il parere è conforme a quello del relatore.

Signora Presidente, come è noto a tutti, c'è grande preoccupazione in Italia, in particolare a Genova e a Castellammare di Stabia, ma anche a Riva Trigoso, per l'annuncio terribile, nei numeri

ancora la questione, e ritengo sia importante che nell'Aula del Senato siano rappresentati il dolore e la preoccupazione che ieri ho visto negli occhi dei lavoratori davanti ai cantieri di Sestri Ponente. Purtroppo, oggi a Genova, come sapete, vi sono stati anche degli scontri. E c'è una tensione terribile in chi non sa se potrà dar da mangiare ai propri figli. figli. Io chiedo che il Governo, che si è detto disponibile, nella persona del ministro Romani, a fare un incontro il 3 giugno, anticipi questo incontro. Non si può rimanere fino al 3 giugno in questo stato di tensione. chiedo che non sia solo il ministro Romani, ma il Governo nel suo insieme, nelle sue massime responsabilità, a prendere in mano questa situazione. Ovviamente, io mi auguro che, intervenendo che, intervenendo anche come azionista di Fincantieri, affermi che siti produttivi non possono essere chiusi e che non possa esserci un taglio occupazionale di queste dimensioni. È una tragedia non solo per i singoli che la stanno vivendo,

Signora Presidente, purtroppo anche io devo evocare in questa Aula i problemi che attanagliano le famiglie italiane che non sono più in grado di sapere se riceveranno lo stipendio del capo famiglia. Voglio parlare della Over Meccanica di Verona, e credo che la collega Bonfrisco possa seguirmi. Io ho presentato una interrogazione urgente, e non avrei sollevato di nuovo il problema se il Governo avesse risposto. Era un'interrogazione urgente, signora Era un'interrogazione urgente, signora Presidente, perché questo nostro Governo si è molto qualificato sulla difesa della italianità. La Over Spa è un'azienda di meccanica fine di grande qualità e tradizione. per difficoltà ad avere crediti. I proprietari si sono fatto carico di garantire la continuità del lavoro, anche mantenendo il numero dei dipendenti. Si erano affacciate due cordate, una tedesca e una francese; quella tedesca si è già ritirata e non abbiamo notizie di cosa accadrà per quella francese. Nell'attesa di trasferire i Ministeri, i Ministri

Se si inventano modalità che invece di essere di aiuto creano difficoltà, mi pare che il Governo possa anche rivedere le sue intenzioni e le sue scelte. *(Applausi

la vicenda di due Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Fondazione Santa Lucia ed il Gruppo San Raffaele. Queste due strutture rappresentano il fiore all'occhiello non solo della sanità del Lazio, ma dell'intero Servizio sanitario nazionale

nell'interesse complessivo del Servizio sanitario nazionale. Non voglio fare differenze fra le due strutture, né tanto meno ricordare cosa fa una e cosa fa l'altra. Il problema di fondo è che in esse sono ricoverati quasi 6.000 cittadini, non solo del Lazio

non solo per la dimensione del problema, cioè per il rischio che, tra lavoratori ed indotto, si determini una ferita

che proprio in quelle aree ha trovato un elemento di riferimento qualitativo di grande importanza e di grande valenza. Ecco perché credo che si tratti di una di quelle vicende che non riguardano un singolo Ministero e che non possono essere affrontate con un tavolo di crisi che si apre sì con puntualità e con grande attenzione, ma che sta dentro la normalità delle vicende e dei rapporti di crisi.

Presidente, stamattina alla Fincantieri di Palermo si è tenuta un'assemblea: circa 2000 lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro. La Fincantieri ha dichiarato che

nell'ex manifattura tabacchi, un deposito che la Fincantieri utilizzava. Questo abbattimento serve soltanto a far vedere il mare agli eventuali clienti di questo albergo a cinque stelle. La verità è che la Fincantieri subirà una stretta dal punto di vista economico e la Fintecna raggiungerà il proprio obiettivo realizzando un albergo a cinque stelle con il mare davanti, e sulla destra le gru della Fincantieri e i relativi rumori provocati dagli abbattitori della stessa struttura.

La volta scorsa il ministro Scajola in quest'Aula raccontò bugie sulla Fiat, che ancora non riapre. Adesso il Ministro aspetterà il 3 giugno per dire ancora bugie. Queste bugie le venga a dire subito e dia garanzie per il futuro dei lavoratori della Fincantieri.

Il Governo non si è solo preoccupato della difesa dell'italianità. In questo caso, ad esempio, di fronte a due cordate, una tedesca e una francese, disponibili all'acquisizione di quest'azienda solo a determinate condizioni, il Governo ha ritenuto di dover difendere innanzi tutto il ruolo dei lavoratori,

dei cospicui finanziamenti alla cassa integrazione: mi riferisco soprattutto a quella in deroga, che abbiamo voluto estendere alle piccole imprese, non concedendo soltanto alle grandi imprese di poter accedere alle forme tradizionali di ammortizzatori sociali, ma consentendo l'accesso anche a quel tessuto delle piccole e medie imprese, vera ossatura del nostro sistema economico, che nel Nord-Est ha una delle sue capitali. L'orgoglio di aver esteso alle aziende artigiane questo sostegno, che per noi vuol dire sostegno al capitale alla nostra risorsa più importante, fa sì che la CGA del Veneto possa oggi segnalarci le disfunzioni che il *click day* ha peraltro generato non a causa delle nostre normative, ma per evidenti motivi di carattere evidenti motivi di carattere burocratico. Sono qua per sostenere, insieme a tutti i parlamentari del nostro territorio, gli sforzi che il Governo sta compiendo per dare risposte adeguate,

si allaccia ad un fatto di attualità; il Senato sta promuovendo l'ulteriore pubblicità della

Signora Presidente, non per essere ripetitivi, ma come Gruppo Lega Nord, vogliamo ribadire la preoccupazione per tutti quei lavoratori e quelle famiglie che in Fincantieri stanno rischiando il posto di lavoro e la busta paga mensile.

in attuazione sulla tracciabilità del rifiuto. Stiamo vivendo dunque un momento particolare, e siamo sicuri che i Ministri preposti si attiveranno per il meglio; confidiamo comunque nella buona volontà di tutte le parti politiche affinché, sedute attorno ad un tavolo, facciano sì che i lavoratori, che mantengono la famiglia e rischiano il loro posto, possano avere certezze per il loro futuro a venire, per Fincantieri, per l'azienda di Verona e per tutte quelle aziende che soffrono un periodo di vera crisi.

e convinta preoccupazione per la situazione che si sta determinando in tutto il Paese, ma soprattutto nell'area di Castellammare di Stabia, per la grave crisi della Fincantieri.

dell'offerta di pari prodotti ad un prezzo nettamente inferiore. Questo non significa però, signora Presidente - e la ringrazio per la condivisione che sento già di recepire da parte sua

Immaginiamo che il Governo, anche attraverso il presidente Berlusconi ed il sottosegretario Letta, riesca ad individuare un percorso che possa riallocare sul mercato del lavoro

possa riferire al presidente Schifani dell'assoluta necessità - ho parlato poco fa con il prefetto di Napoli e con i sindaci della penisola sorrentina

la società Fincantieri. Questa è una crisi preannunziata, ma che non si può risolvere in modo così brutale, perché le proteste dei lavoratori coinvolgono uno

che il Governo dovrà tenere a breve per rasserenare le famiglie e contribuire a trovare soluzioni idonee affinché non ci siano azioni